Discussione del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Devo esprimere innanzitutto un ringraziamento e un riconoscimento a tutti i componenti della 5[a] Commissione, che si stanno impegnando in maniera molto forte, in particolare ai Gruppi di opposizione, che hanno scelto un atteggiamento assolutamente responsabile e collaborativo. Siamo ad un buon punto del nostro lavoro: posso dire così. Dei tre grandi fascicoli

l'attenzione della Commissione, due sono stati completati. Abbiamo però bisogno, signor Presidente, ancora di qualche ora di tempo per poter completare il nostro lavoro. Quindi sarei qui a chiederle di poter utilizzare ancora tutta la giornata di domani per i lavori della Commissione e quindi di poter arrivare in Alla luce di quanto comunicato dal presidente Tonini, l’esame in Assemblea del disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2018 avrà luogo mercoledì 29 novembre, dalle ore 9,30 e - se necessario - nella successiva seduta di giovedì 30 novembre, con inizio sempre alle ore 9,30, salvo successive determinazioni.